per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti», premesso che: a partire dal 1º gennaio

La seduta è ripresa. Prego i colleghi

che il sostegno alla richiesta di voto elettronico sugli emendamenti riferiti ad un determinato articolo si intenderà estesa anche agli emendamenti improcedibili, ove ne venga richiesta la votazione: è un modo per semplificare nel caso di emendamenti

chiedo che l'emendamento venga preso in seria considerazione da chi ritiene di dover far qualcosa per i giovani che si offrono all'importante professione del giornalista e poi vengono mortificati da condizioni di lavoro umilianti pressoché in tutta Italia, ma in particolare in alcuni contesti. Sappiamo tutti cosa sia il precariato, ma

e superano *test* di accesso a scuole più o meno prestigiose, che poi vengono costretti dalle cosiddette condizioni di mercato a vendersi - di questo si tratta

di questa importante funzione, prima ancora che professione. A noi questo sembra il minimo sindacale

una disanima preliminare rispetto ai ricorsi giurisdizionali delle querele e richieste risarcitorie temerarie. Ne abbiamo parlato con il Sottosegretario, che ha dimostrato una sensibilità sul punto, ma purtroppo l'emendamento non è stato accolto. In una fase in cui, a seguito dell'afflusso della domanda di giustizia a una magistratura ordinaria purtroppo non in grado di risolvere in maniera sufficientemente efficiente e veloce il contenzioso, interporre degli organi a valenza extragiudiziale (comunque con una natura persuasiva, etica, non vincolante, ma fortemente significativa per la categoria che la rappresenta) che siano in grado di rappresentare una deflazione del contenzioso stesso. Ciò ha una doppia valenza: da un lato quella di dimostrare alla categoria

in maniera non pretestuosa uno strumento importante qual è quello dell'informazione; dall'altro, naturalmente (e il dato non è irrilevante)

Oltretutto - e questo lo abbiamo fatto presente al Sottosegretario e ci dispiace che non sia stato sensibile sul punto - questa è una tradizione che non abbiamo inventato noi, anzi è una tradizione a cui ci siamo avvicinati troppo tardi. I modelli extragiudiziali non vincolanti di composizione delle controversie, in un'ottica anche etica e deontologica di autodisciplina della categoria, in altri ordinamenti (certamente nell'ordinamento anglosassone e in quello americano, ma anche in altri ordinamenti europei molto contigui al nostro), esistono dagli anni '70. Esistono ed hanno un forte successo, non solamente rispetto alla categoria stessa, ma anche agli occhi di tutti coloro che alla categoria si avvicinano, ingenerando un rapporto mutuamente fiduciario: la categoria si autodisciplina e coloro i quali accedono allo strumento dell'informazione

che oltretutto vanno nella direzione di quanto il Governo dice di voler fare, cioè potenziare e valorizzare - l'ho sentito dire tante volte dal ministro Orlando - modelli extragiudiziali di composizione delle controversie, in sede di autodisciplina e di autocontrollo deontologico della categoria; però poi, all'atto pratico e allo stato dei fatti, quando ci si trova al momento di applicarli concretamente non lo si fa. E questo francamente ci dispiace.

previsione di una riduzione per le imprese che superano, nei confronti del proprio personale, dei propri collaboratori e amministratori, il limite massimo retributivo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno

Grazie,

la riduzione non è quantificata, neanche in un arco discrezionale. È una riduzione indiscriminata, che potrebbe andare

nei confronti del proprio personale e dei propri collaboratori e amministratori, esiste un limite massimo retributivo. Mi pare che ci sia ancora da chiarire la portata di questo emendamento, perché l'eccessiva discrezionalità lasciata a chi poi deve attuare la norma potrebbe vanificare l'intento di queste proposte emendative.

Se è vero, come è vero (o in parte), che il settore interessa la libertà di informazione, credo - come giustamente ha detto prima il senatore D'Alì che la previsione di una riduzione debba essere accompagnata, fin dalla delega, dall'individuazione dei criteri oggettivi in virtù dei quali la riduzione stessa deve essere fatta. In caso contrario, daremmo al legislatore delegato una sorta di delega in bianco, per la totale assenza di criteri, in una materia garantita sotto il profilo costituzionale. Pur non essendovi - come diceva prima sempre il senatore D'Alì - alcuna contrarietà in ordine a questo emendamento, credo che un ulteriore approfondimento dello stesso, con l'individuazione di una maggiore specificazione dei criteri in virtù dei quali operare la riduzione, possa essere senz'altro utile.

Grazie, ai propri dipendenti, consulenti e amministratori retribuzioni esorbitanti, che si scaricano, poi, sui cittadini, dal momento che esse vanno ad incidere sui costi. Dobbiamo accollarci noi quei costi? Poiché il Governo ha sbandierato di voler mettere un tetto alle retribuzioni nella pubblica amministrazione, quando abbiamo a che fare con imprese che ricevono contributi statali dobbiamo Il testo era chiaro: se dai retribuzioni d'oro, non hai diritto a contributi. E questo era condivisibile e chiaro anche ai cittadini che ci ascoltano da casa. Su quel testo Governo e relatore si erano rimessi all'Assemblea, nel caso non fosse stata accettata la proposta di conversione in ordine del giorno. Un ordine del giorno in una legge delega a me fa veramente ribrezzo

noi abbiamo aperto la strada a una beffa, a una farsa. Si dica dimezzamento, si dica riduzione dell'80 per cento, si dica riduzione pari

di una finalità importante ed *erga omnes*, non legata solamente alle imprese editoriali o al senso stretto del provvedimento in esame. Il senso è lato ed è quello di garantire ai cittadini la possibilità di conoscere quali sono gli interessi.

Grazie,

linea di demarcazione - ripeto che deve essere netta e non evanescente - tra il conflitto e la rappresentanza di interessi. Ed è questo il motivo per cui riteniamo che un registro delle imprese operanti nel settore della Grazie,

spesso nel Consiglio nazionale sono state poste all'ordine del giorno tematiche riguardanti i praticanti pubblicisti e professionisti che, pur prestando la loro opera presso imprese editrici che fruivano di significativi contributi statali, non avevano poi percepito i compensi dichiarati dalla proprietà per accedere al finanziamento stesso. L'emendamento 3.303 consentirebbe di accertare

esperienze imprenditoriali che hanno come unico obiettivo gestire e manipolare l'informazione: attraverso il controllo dell'informazione, il potere condiziona la cosiddetta opinione pubblica. defunte. È arrivato qualcuno, cioè lo Stato italiano, che ha detto: «Lazzaro, alzati e cammina», e un giornale a caso, «l'Unità», ha ripreso a editare, ma è uno tra i tanti. A nostro avviso, tutto il rispetto nei confronti di forme di attività economica rispettabili in altri casi non va portato, perché altrimenti dovremmo

ribadendo come il *web* sia la dimensione all'interno della quale con assoluta libertà tutti possono fare informazione, chiedo all'Assemblea di poter quantomeno ridurre l'entità dei finanziamenti, a meno che non ci si voglia ritenere all'altezza di Gesù Cristo e far risuscitare anche i morti.

Mi chiedo se esista effettivamente una parificazione tra imprese nel nostro Paese e mi pare che le imprese editoriali siano imprese. A qualsiasi altra impresa di altra natura che debba partecipare a una gara con il settore pubblico - non si parla di ricevere contributi - viene chiesto il famoso documento unico di regolarità contributiva caso parliamo non di partecipare a una gara, ma addirittura di ricevere un contributo pubblico e non vogliamo prevedere che sia esibita eguale certificazione?

addirittura di percepire un contributo statale e non si vuole prescrivere che queste imprese esibiscano un documento che certifichi la regolarità stipendiale e contributiva?

Grazie,

è già nei principi generali della legge. Ma un'ulteriore specificazione sarebbe opportuna. Credo occorra fare una piccola riflessione su questi principi.

sulla formulazione del comma 7*-bis*, dove viene precisato che: «All'atto dei pagamenti, l'impresa deve essere in regola con le attestazioni rilasciate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con i versamenti dei contributi previdenziali e non deve risultare inadempiente in esito alla verifica di cui all'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602». A me pare che il punto che viene sollevato sia già previsto nella norma che andiamo ad approvare.

mi permetto di reiterare la richiesta, perché sarebbe come dire che la previsione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che è generica e non di carattere contabile (è semplicemente una verifica), applicata in termini generali renderebbe inutile un documento di regolarità contributiva, che è ciò che noi chiediamo in questo caso. E non lo chiediamo in maniera peregrina. Lo chiediamo perché al Consiglio dell'ordine sono pervenute numerose segnalazioni da parte di giornalisti, praticanti pubblicisti e professionisti, che, pur avendo prestato la loro opera presso imprese editrici che usufruivano di contributi statali, non hanno percepito i compensi dichiarati dalla proprietà per accedere al finanziamento. Pertanto, collega relatore, noi chiediamo qualcosa in più.

Prevediamo un provvedimento, su cui insistiamo con il relatore e con il sottosegretario Giacomelli, che abbia la stessa valenza e la stessa capacità di controllo pervasivo che ha il documento di regolarità contributiva (DURC).

ringrazio il relatore per la possibilità offerta e per aver valutato positivamente l'intento dell'emendamento.

il libero pensiero e il libero esercizio del pensiero su Internet, e non quello, eventuale e potenziale, di allargare la platea dei fruitori e *g)* si corre il rischio che la platea dei fruitori del finanziamento pubblico, esteso anche ai quotidiani *online*, si estenda anche alle due voci che verrebbero escluse da questo emendamento, che sarebbero

una versione telematica di una testata cartacea, potrebbe acquisire la definizione di quotidiano *online* e, quindi, una indipendente possibilità di accedere ad ulteriori finanziamenti pubblici.

Grazie,

se non dovessero essere approvati i punti che lui ha sostenuto, almeno cominceremmo ad avere un minimo di regolamentazione su una situazione

Grazie,

che il Governo valuti l'opportunità di definire i quotidiani *online* con tutte le caratteristiche che ho appena indicato.

chiederei di formulare in termini tali da poter svolgere un approfondimento. La questione che solleva il senatore Crimi è reale e gliene do volentieri atto.

sull'ordine del giorno. Io credo si sia persa un'occasione importante, quanto sostenuto dall'emendamento Crimi va nella direzione giusta, perché si sente assolutamente la mancanza di una regolamentazione di tutto quello che va *online*. in un giornale (anche cartaceo) sa bene che non è mai possibile fare una pubblicazione integrale di contenuti originali, perché si prendono le agenzie di stampa e si mettono *online* i comunicati. Non è mai possibile non lo era neanche ai tempi d'oro del giornalismo, quando le redazioni erano piene di giornalisti. Ora, con l'attuale crisi occupazionale, si è costretti a mettere

Signor Presidente, riprendendo la linea che il relatore ha già esposto e che io condivido, vorrei provare a interloquire con il senatore Crimi. Anche io trovo, come ha appena detto il senatore Mazzoni, che questa sia una occasione importante. Tuttavia, nel merito dei due punti specifici di cui il relatore ha chiesto la soppressione, non so se sia possibile immaginare una versione di un quotidiano *online* interamente autonoma da un punto di vista editoriale e se ciò finirebbe per escludere totalmente ogni possibilità. Se, invece, ci fosse la possibilità di dire che il quotidiano *online* non può essere l'integrale, automatica e esclusiva trasposizione in rete di un quotidiano cartaceo, questo è già un concetto sul quale io mi troverei

notizie, nella mia esperienza (e io vengo politicamente dal "Vecchio Testamento"), ricordo una specie di quotidiano, di attività, che raccoglieva esattamente articoli e notizie relative a un certo filone culturale.

è attività di raccolta di articoli, di agenzie e di notizie ha questa natura indeterminata, casuale o meramente tecnologica; può esservi benissimo una iniziativa editoriale

oggi, per la verità, più che preoccuparci dell'assemblaggio dei lanci di agenzia, bisogna preoccuparci dell'influenza che i *post* su Facebook o su altri *social* hanno sui giornali. Ormai,

complessivamente, come intuizione, condivisibile. Mi piacerebbe sapere se lei ritenga vi sia la possibilità di una determinazione nel merito

definisce l'equo compenso. Ricordiamo da dove nasce questa misura. Essa è contenuta nella legge 31 dicembre 2012, n. 233, che stabilisce che i compensi dei giornalisti non titolari di un contratto di lavoro subordinato devono essere parametrati a quelli dei colleghi titolari di un contratto subordinato. Inoltre, la legge prevedeva che venisse istituito un registro delle

Quali sono i rischi di una commissione che questo provvedimento

Ci troveremmo così a dover intervenire in un secondo momento e avere quella situazione di precarietà, che tanto piace al Governo delle mille proroghe, ma che non è compatibile con la trasparenza e l'affidamento alla legge da parte del cittadino. Abbiamo così due conseguenze pratiche. Da un lato, l'impossibilità di adeguare questo giusto compenso dei giornalisti e il perpetrarsi di quelle situazioni di sfruttamento dall'altro, il fatto che se l'elenco degli editori virtuosi rimane fissato una volta per tutte, quelli che nel frattempo potrebbero realizzare la convenienza ad adeguarsi a questi principi, a vantaggio della categoria dei giornalisti, non avrebbero più questo incentivo (cosa fatta, capo ha), mentre chi risulta iscritto potrebbe tranquillamente poi modificare la propria *policy* perché nessuno avrebbe più titolo per aggiornare questo elenco. Noi chiediamo semplicemente che, ogni due anni, la commissione continui a tenere aggiornati l'elenco degli editori virtuosi e l'equo compenso per i giornalisti. La legge è senza

forse sarebbe più opportuna una breve interruzione, altrimenti il collega Crimi non potrà partecipare ai lavori né votare. Trattandosi di qualche minuto probabilmente non sarebbe neanche impattante sui lavori dell'Aula.

Grazie, chi esercita abusivamente l'attività di giornalista venga incriminato ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.

si conclude poi con un arroccamento corporativo qual è la previsione di sanzioni penali per l'esercizio abusivo della professione. che tentativi di addebitare il reato di cui all'articolo 348 del codice penale, esercizio abusivo di una professione, ai giornalisti non iscritti all'albo ci sono stati solo negli anni Sessanta ma si sono conclusi con una sentenza della Corte di cassazione del 1971 che ha sottolineato la difficoltà di applicare l'incriminazione rispetto ad una attività che è comunque segnata dal principio di libertà di manifestazione del pensiero. Da allora nella giurisprudenza non si trovano più tracce, nei repertori, di procedimenti penali a carico di giornalisti cosiddetti abusivi. Un'ultima considerazione, Presidente: per la professione giornalistica, come sa bene il sottosegretario Giacomelli, la legge ordinamentale del 1963 prevede la possibilità di conseguire l'iscrizione all'elenco dei pubblicisti per coloro che possono dimostrare di avere svolto un'attività non occasionale e retribuita da almeno un biennio per testate regolarmente registrate. Ora, questa è una modalità di accesso della quale il legislatore, e quindi noi, dovremmo tenere conto, perché chiunque non sia ancora iscritto all'albo dei pubblicisti e scriva per un giornale per ottenere la tessera di pubblicista rischia di essere incriminato. Io credo che questa sia una norma illiberale che dovrebbe essere espunta da questo provvedimento.

L'emendamento 5.3 prevede l'impossibilità di essere iscritti all'albo per i politici o gli appartenenti alle organizzazioni sindacali che hanno rivestito tali incarichi nei tre anni precedenti. Questa è una misura di trasparenza. È difficile immaginare che un politico che prima rappresentava ragioni di parte poi, improvvisamente, possa essere credibile nel rappresentare i fatti in maniera oggettiva. A parte questo, dobbiamo anche evitare come di incorrere in un conflitto di interessi. È stata infatti votata da quest'Assemblea una riforma che riduce il numero dei senatori, e per quanto ci riguarda lo riduce totalmente, perché noi non siamo e non saremo nell'immediato consiglieri regionali per cui ci troveremo ad essere serenamente disoccupati. Non vorrei che ci trovassimo di fronte una serie di provvedimenti che consentano o addirittura istituiscano le carriere successive alle persone che hanno votato questa riforma. Faccio un esempio: nella legge sulla normativa del lobbismo, cioè dell'attività di di rappresentanza di interessi, si prevede l'istituzione di una sorta di patentino per chi svolge questa attività. Ebbene, in quella legge è previsto un periodo di "raffreddamento": se si è fatto il parlamentare fino a ieri, si deve aspettare un po' prima di andare a fare il lobbista che preme sui parlamentari. E così dovrebbe essere nel campo del giornalismo: dovrebbe esserci un periodo di raffreddamento, di pausa e di *vacatio*. Noi lo individuiamo nei tre anni. Rappresentiamo pertanto all'Assemblea l'opportunità di evitare di essere considerati in conflitto di interessi votando contro questo emendamento

dichiarato spesso anche dal *Premier*, occorre togliere il più possibile il controllo degli organi di informazione e soprattutto anche degli organi di controllo e di gestione dell'informazione come, per esempio,

almeno di lasciare del tempo o comunque limitare il passaggio rapido dalla politica all'ordine dei giornalisti, alle organizzazioni sindacali o alle segreterie. Questo semplicemente per evitare che i partiti gestiscano direttamente l'informazione. Mi rendo conto che non avendolo votato nella legge sulla *governance* della RAI, non lo farete neanche in questa, ribadisco però la discrasia, la lontananza,

penoso della libertà d'informazione in Italia e l'assoluto silenzio di quest'Aula ogni volta che ci si pone tali questioni.

Comaroli, mentre lei interviene, prego i senatori Segretari di disporre l'estrazione delle schede perché vedo molte schede in posti non occupati per evitare equivoci

noi abbiamo presentato due emendamenti sul tema molto delicato e serio della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo.

intercorre tra il vecchio contratto, quindi la vecchia convenzione, e quello nuovo disposto attraverso il nuovo affidamento.

noi vogliamo parlare di privatizzazione della RAI, di abolizione del canone con proposte alternative di finanziamento (consapevoli che l'articolo 81 della Costituzione non può essere saltato a piè pari

apparecchi e supporti per la ricezione e la decodificazione del segnale pubblico. 6-*bis*.303 avanziamo un'altra proposta volta alla privatizzazione della RAI, imponendo a tutte le televisioni private di trasmettere una parte di programmazione di servizio pubblico, cosa che peraltro già fanno,

molto più plurale di quello che offre la RAI. Per cui passare in maniera strutturale un po' di servizio pubblico alle emittenti locali sarebbe opportuno. Come? Eliminando nel contempo il canone e disponendo che questi programmi pubblici siano finanziati attraverso i ricavi pubblicitari che l'emittente ottiene dalla vendita degli *spot* e dei programmi stessi.

abbiamo constatato parlando con i nostri cittadini negli ultimi mesi sulla questione del canone,

andiamo a criptare tutti gli altri programmi che non sono definiti tali. A questo punto, paga il canone chi mette il *decoder*, anche nel servizio pubblico, e noi invece andiamo a garantire il servizio pubblico per tutti, in maniera aperta

se qualcuno mi impone di pagare l'abbonamento, allora è una tassa. Per cui l'abbonamento non esiste: è la tassa della RAI, perché l'abbonamento è un'altra cosa a casa mia.

E come andiamo a finanziarlo? Qui sta la chiave di volta, perché prendiamo due piccioni con una fava: aboliamo il canone RAI e andiamo a finanziarlo con la legalizzazione della prostituzione.

vada alle Regioni, in conformità alla normativa sul federalismo fiscale per le televisioni locali. È chiaro che questa sembri una utopia, ma con lo scenario che si presenta ai nostri occhi nostri occhi anche molti colleghi del PD stanno rimpiangendo quella riforma costituzionale proposta dall'allora ministro Calderoli, con la quale si prevedeva anche di andare a rivedere tutte le tutte le questioni riguardanti l'informazione, immaginando di demandare alla periferia, cioè all'ente locale, le risorse e la gestione pure del servizio pubblico locale.

Di questi, 165 sono quelli finalizzati in parte al fondo e in parte alle agevolazioni fiscali. È evidente, però, che ne restano 335 che vanno al concessionario radiotelevisivo.

a rivolgersi a questo unico soggetto. Io non posso però dimenticare tutte le polemiche nate nei mesi scorsi, e adesso un po' attenuatesi, rispetto agli stipendi di coloro che svolgono funzioni di amministrazione o di giornalismo all'interno del sistema della RAI.

ai dirigenti e ai dipendenti (...) non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000». Vi era la previsione che questo limite interessasse le società direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni dello Stato sia da altre amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati.

Cosa accadde? Giustamente in questo caso, il Governo Renzi anticipò l'entrata in vigore, anziché a maggio 2016, a maggio 2014 e, a un anno di distanza (finalmente, si può dire), nel giugno 2015, il consiglio di amministrazione della RAI aveva deliberato che a tutta l'azienda si applicasse il tetto fissato dalla legge per la pubblica amministrazione, cosa assolutamente sacrosanta perché è una legge dello Stato. Ma era il consiglio uscente. Dopo pochi giorni il nuovo consiglio ha ha avviato il collocamento di 350 milioni di *bond*. È chiaro che le quotazioni azionarie e i *bond* non c'entrano assolutamente nulla: è stato il trucco con cui aggirare l'ostacolo; conseguentemente a questo trucco, il giorno dopo gli stipendi hanno ripreso a salire. Ricordo a me stesso e all'Assemblea il direttore generale Campo Dall'Orto, che si vede garantiti 650.000 euro

da quel decreto-legge e che non stanno neanche lavorando. Per quanto mi riguarda, è una vera vergogna che vi siano soggetti che da anni percepiscono 300.000 euro per non fare assolutamente niente*.

Nel nostro emendamento vi è la previsione del rinnovo della convenzione; ci sarà uno schema

che applichi i limiti stipendiali che si applicano a tutta la pubblica amministrazione *(Applausi del senatore Candiani)*, indipendentemente dal fatto che lo stesso soggetto abbia quotato dei *bond*, perché si è trattato di un trucco per aggirare il il tetto stipendiale. È una questione di giustizia e di equità; l'abbiamo parzialmente introdotta rispetto a tutti i soggetti che riceveranno dei soldi pubblici per editare, mi sembra ancor più obbligatorio rispetto a un concessionario che assumerà la concessione

Questo problema è stato discusso in Commissione parlamentare di vigilanza RAI e abbiamo votato all'unanimità. Colleghi del Partito Democratico, voi avete

Sperequazioni, stipendi diversi: ci sono delle stratificazioni. Dopo di che, siccome viviamo in un'epoca di trasparenza (un po' sospesa al Comune di Roma negli ultimi tempi, ma tendenzialmente viviamo in un'era di trasparenza),

dopodiché non si guasta niente: con 240.000 si campa lo stesso. Noi siamo la casta, ne prendiamo di meno e siamo dei privilegiati, io me ne rendo conto, rispetto alla massa dei cittadini. ben consapevole di questo e dobbiamo sicuramente fare di più per ridurli. Poi chi guadagnava zero e ora guadagna 5.000 e fa la parte dell'eroe è passato da zero a 5.000, ma lasciamo perdere anche se anche in questo caso ci sarebbe da fare una discussione spinosa. Approviamo dunque questi emendamenti in coerenza

1.582.000 famiglie in povertà assoluta. Sono 4.598.000 persone secondo il rapporto ISTAT e nel Mezzogiorno quattro famiglie su dieci sono in condizioni di povertà relativa. milioni di persone hanno difficoltà ad accedere alle cure, però anche i poveri pagano le imposte, per esempio il canone RAI per cui è prevista, è bene dirlo, un'esenzione

per la salute? Bene, questo è come il Governo ricompensa i cittadini che - poveri - si tolgono il sangue obbligatoriamente per pagare il canone RAI, garantendo ai dirigenti stipendi da 600.000 euro l'anno, come al direttore generale Campo Dall'Orto. Come mai così tanto? Come mai così tanto, se è stata fissata una norma per i dirigenti pubblici con un tetto a 240.000 euro? Ad inizio 2014 veniva fissato questo tetto, però con una il tetto non vale per le società che emettono titoli negoziati su mercati regolamentati.

Siamo arrivati allo scandalo degli stipendi d'oro perché poi, a maggio 2015, è arrivato il via libera del consiglio di amministrazione RAI all'emissione di quelle obbligazioni. Prima il tetto vigeva, poi non più. Questo lo denunciava un esponente del Partito Democratico, Michele Anzaldi, che strepitava dicendo che è scandaloso e di cattivo gusto, in questo momento molto difficile per il Paese, che la RAI non abbia trovato un minuto per rassicurare gli italiani che il tetto agli stipendi dei dirigenti non sarà aggirato. Si arriva ad ottobre 2015 e, puntualmente, si vota la legge di riforma della *governance* RAI e quando il Movimento 5 Stelle dice di togliere quella postilla dal sapore vagamente truffaldino, tutto il Partito Democratico vota contro, salvo poi battersi il petto quando lo scandalo esplode. Nel luglio 2016 infatti, poco tempo fa, emergono le indiscrezioni sui mega stipendi. allora al momento di chiudere questa saga, questa farsa che suscita sdegno nei cittadini e porta vergogna alle istituzioni. Dobbiamo semplicemente ripristinare questo tetto anche per la RAI e per tutte le società. Dobbiamo togliere questo distinguo.

Antonio Campo Dall'Orto è stato scelto e assunto da Renzi, forse questo è il motivo che spiega come mai gli vengono garantiti 600.000 euro. Forse il motivo lo vediamo anche nei palinsesti, nel minutaggio che viene dato alle istanze, per esempio, per il no al *referendum* costituzionale invece che al sì. Lo abbiamo visto già in precedenza su come è stato trattato il tema del *referendum* contro le trivellazioni in mare. quando si è votata la legge di riforma della *governance* RAI, 257 parlamentari, cioè la stragrande maggioranza del PD, si sono presi la responsabilità di mantenere quel cavillo,

O noi togliamo oggi quel cavillo ed eliminiamo la norma secondo cui emettendo obbligazioni si può aggirare il tetto oppure chiediamo ai parlamentari del Partito Democratico di decurtarsi lo stipendio. Non si vive male, come ha detto poco fa il collega Gasparri, con 240.000 euro. Si vive benino. Ebbene, si vive benino anche con i nostri stipendi, anche se per un motivo di coscienza, intendiamo restituire ai cittadini almeno le conseguenze delle nostre azioni. Mi si dirà che è poca cosa perché, se andiamo a vedere quanto costa un politico per le scelte

tempo 1) si applica con anticipo il tetto agli stipendi; tempo 2) viene formulata un'emissione di *bond*; tempo 3) il campo di esclusione, perché si perfeziona la fattispecie delle società emittenti strumenti finanziari quotati. Credo che per qualificare ciò che è successo

Ho memoria di posizioni attive della RAI e poi di progressivamente indebitamento, ma fatto per linee bancarie e non per emissione di titoli. luogo, se non ho cattiva informazione, l'importo dell'emissione è assolutamente elevato. Credo siano 400 milioni, che sono un'emissione di enorme rilievo per un soggetto che non ne ha mai fatte. Inoltre, dovrebbe essere noto in questa sede il costo di quella emissione in termini di interessi, il costo delle commissioni per piazzare quei titoli infine, la gestione successiva di quella posizione finanziaria. la dimensione di costo dell'operazione (evidentemente strumentale), i particolari vantaggi tratti da quella emissione e fondamentalmente - forse non per questa sede, ma per altre, importanti - il danno erariale.

dovrebbe portare a un'attenta riflessione su un fenomeno non solo dilagante ma oramai costante, che anche in questo caso specifico dev'essere chiamato femminicidio. Tiziana, la cui rovinosa vicenda, ossia la circolazione dei filmati *hard* diventati virali sul *web*, non necessita in questa sede di essere ripercorsa, è stata di fatto però impossibilitata a condurre un'esistenza dignitosa. L'interruzione di tutti i rapporti sociali, la vergogna, lo stato di depressione, il primo tentativo di suicidio, un peso insostenibile, una morte annunciata e quindi anche prevedibile: una violazione della *privacy*, una violazione a tutti gli effetti che l'ha costretta a cambiare dapprima identità e poi a rivolgersi alle competenti autorità al fine di ottenere ristoro e giustizia nei confronti di chi ha reso pubbliche le immagini, quanto dei *social* responsabili anch'essi di aver diffuso il video in questione. Mi riferisco ai vari *social* come Facebook, Yahoo, Google e YouTube. Il giudice incaricato del caso in esame ha riconosciuto la lesione del diritto alla *privacy* della donna, contestando nello specifico ai *social* la non immediata rimozione dei contenuti lesivi della reputazione. Ma questo non può bastare, ovviamente. Ebbene, i contenitori *web* non posso racchiudere e veicolare ogni tipo di dato, senza apporre quei filtri che tutelano la dimensione umana. Occorre tenere ben presente che la libertà di ognuno termina laddove comincia quella altrui. Bisogna trasmettere l'importanza delle relazioni umane. È necessario a tal fine far comprendere come il sostrato delle relazioni sia necessariamente il rispetto della vita altrui. Vi deve essere una cabina di regia che coinvolga, nei casi analoghi, simili o similari a quello di cui si sta discutendo, anche i contenitori e diffusori presenti sul *web*. La cabina di regia sul territorio deve ricomprendere servizi come la sanità e l'area della giustizia, ma *in primis* anche le misure necessarie per promuovere i cambiamenti e quei comportamenti socioculturali delle donne e degli uomini. I dati sul fenomeno del femminicidio sono sconcertanti, come sappiamo: le le donne morte negli anni sono più di 2.000, eppure la livellazione di statistiche ufficiali non registra il fenomeno del femminicidio che passa anche attraverso il *web*. Occorre comprendere nel dettaglio come la società affronta e vive il fenomeno della violenza di genere contro le donne e quali misure e investimenti adottare in termini di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e ancora quanto e come, a fronte dei sopracitati investimenti, gli italiani percepiscono il fenomeno della violenza di genere e sono liberi da stereotipi e pregiudizi che costituiscono fattori di rischio della violenza stessa. Gli uomini e i ragazzi devono essere resi consapevoli dell'importanza del ruolo e conseguentemente devono essere posti in prima linea nella lotta alla violenza contro le donne come attori principali del necessario cambiamento culturale. Ribadisco anche in questa sede la necessità di avviare un intervento strategico che renda responsabili i politici più consapevoli dell'importanza e dell'efficacia della prevenzione e che renda maggiormente evidente la portata di un fenomeno nella sua dimensione sociale. Per la sua matrice culturale, la violenza sulle donne non può essere contrastata prescindendo da un'analisi di ciò che muove la nostra società. La violenza contro le donne è percepita come un fenomeno diffuso e in aumento, ma che resta ancora una questione relativa alla sfera privata, non emerge nella sua dimensione pubblica e totale. *(Applausi dai Gruppi PD e Misto)*. PRESIDENTE. La Presidenza si associa al cordoglio per la morte drammatica di questa ragazza.

una staffetta con cui, assieme a tante senatrici e tanti senatori, ricordiamo ogni donna che viene uccisa per mano di un uomo a cui è o è stata legata da relazione amorosa. Lo faremo fino a che sarà necessario ricordare al Parlamento e al nostro Paese l'urgenza di arginare la violenza nei confronti delle donne. Nell'intervento di oggi dobbiamo ricordare quattro donne uccise, che si aggiungono alle dieci che abbiamo ricordato dal 30 giugno, quando questa staffetta ha avuto inizio. A Parma, il 10 settembre, Elisa Pavarani, di trentanove anni, è stata uccisa a coltellate; per l'omicidio è stato arrestato ed è indagato l'ex fidanzato. Mi si lasci poi aggiungere a questo episodio il ricordo Michelle Campos Verde, 20 anni, assassinata tre anni fa, purtroppo sempre a Parma, dall'ex fidanzato: la madre era oggi in Senato per la legge sulla cittadinanza. Il 29 agosto a Seregno, in provincia di Monza, Carmela Aparo di 64 anni è stata uccisa a colpi di pistola dal suo compagno. Sempre il 29 agosto a Caramagna Piemonte, in provincia di Cuneo, è stata uccisa a coltellate Pashke Babaj. Il marito è stato fermato per omicidio. L'ISTAT ci informa che in Italia ogni 2,2 giorni viene uccisa una donna; il 46,3 per cento delle donne muore per mano del *partner*. La gravità delle violenze sessuali e fisiche è aumentata. Sono in crescita anche i casi di violenza assistita. Il femminicidio è quasi sempre l'estremo risultato di una serie di comportamenti violenti di lunga data vorrei aggiungere che si inserisce in un contesto sociale che troppo spesso è troppo violento, troppo caratterizzato da un confronto che si basa sull'odio e sulla contrapposizione anziché sulla capacità di confronto e sul rispetto delle persone. Il femminicidio è quasi sempre l'estremo risultato di una serie di comportamenti violenti di lunga data. Con la legge n. 119 del 2013 di contrasto alla violenza di genere, che questo Parlamento ha approvato in attuazione della Convenzione di Istanbul, il nostro Paese ha riconosciuto la violenza sulle donne come violazione dei diritti umani e discriminazione di genere; ha riconosciuto che la violenza sulle donne è un fenomeno sociale che ha le proprie radici nella relazione di potere asimmetrica fra uomini e donne. Per questo la si può prevenire, intervenendo sui fattori che la determinano. Per questo è stato proposto ed approvato un piano contro la violenza sulle donne e, nel frattempo, sono stati rafforzati strumenti di protezione per garantire maggiore sicurezza alle donne minacciate. Bisogna però monitorare che queste misure funzionino e che il piano sia attuato. Per questo abbiamo accolto con favore la notizia che l'8 settembre

Riproponiamo infine con convinzione il nostro appello, un appello alla Ministra per le Pari Opportunità e al Governo tutto: la cabina di regia monitori l'applicazione, i pregi e i limiti della legge n. 119 del 2013 e soprattutto dia piena ed accurata attuazione al Piano contro la violenza. Un appello rivolgiamo ai *media*: si smetta di giustificare gli assassini e di colpevolizzare le donne. Un appello a tutto il Paese, agli uomini e alle donne: sono 160 le donne uccise ogni anno, non possiamo più accettare questa mattanza. Grazie, senatore Pagliari. Sono numeri e vicende impressionanti: io credo si debba continuare nel senso che lei diceva e suggerirei anche delle iniziative molto forti nella scuola, perché è da lì che io credo si debba cominciare per cambiare la cultura degli uomini e delle donne.

Ora, l'invasione di campo di sua eccellenza l'ambasciatore americano in Italia, che pensa di spiegare agli italiani come devono votare, unita a questo fatto, rende particolarmente opportuno che il Governo risponda. Ricordo che tutti i governi del mondo enti territoriali italiani rispondono alle interrogazioni. Solo il Governo italiano risponde solo ad alcune interrogazioni e solo questo Governo ha ulteriormente ridotto il numero di interrogazioni alle quali risponde, per di più scegliendole in modo spudorato solo tra quelle che gli fanno comodo.

in questo momento di rapporti particolarmente intensi tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America (che mi auguro siano sempre più intensi, ma rispettosi della rispettiva indipendenza), il Ministero dell'ambiente spieghi perché ha dato più di 100.000 euro alla Fondazione che si chiama Bill, Hillary and Chelsea Clinton Foundation, che guarda caso ha una certa influenza sul Governo degli Stati Uniti, per cui mi sembra che questo *do ut des* non vada molto bene. Ci vuole trasparenza. Il Ministero dell'ambiente non può usare i soldi suoi. Se il Ministro dell'ambiente vuole dare soldi alla signora Clinton è libero di farlo; non alla sua campagna elettorale, perché è vietato dalla legge degli Stati Uniti, ma alla sua fondazione lo può fare. fa come Ministero, deve per lo meno renderlo noto. Questa omertà è inaccettabile ed è una totale mancanza di rispetto per il Parlamento e per gli italiani. Non vuole rispondere in Parlamento? Vada a «Porta a Porta» a spiegarlo, visto che il signor Presidente del Consiglio umilia il Parlamento e fa le comunicazioni che dovrebbe fare in Parlamento nelle trasmissioni televisive.

sanità è veramente paradossale. Purtroppo, torniamo a immagini pirandelliane, nell'accezione più deteriore, che alcune volte comprimono la possibilità di sviluppo, di ordine e di prospettiva serena cui avrebbe diritto il popolo

esplode la tensione perché le prime carte di questa sorta di atto carbonaro iniziano a girare, con una mortificazione incredibili di territori e anche di grandi realtà

potevano causare ostilità da un punto di vista del consenso elettorale, si affretta a dichiarare che la Sicilia non ha presentato alcun atto di rimodulazione della rete ospedaliera e che, piuttosto, è il Governo centrale ad aver evidentemente falsa), una condizione in virtù della quale la Sicilia è costretta ad accettare questo piano. La verità è che, purtroppo, se non fosse drammatico, sarebbe esilarante osservare che,

che l'invito da me esteso ai parlamentari di tutti i Gruppi di occuparsi della Sicilia e della sanità possa essere accolto, al di là delle posizioni politiche di ciascuno. **Per

Grazie,